Signor Presidente, onorevoli senatori, stiamo affrontando con tutti gli strumenti a disposizione la questione relativa alla diffusione nel nostro territorio dell'organismo nocivo da quarantena *popillia japonica*. Nel nostro Paese la presenza di *popillia japonica* è stata segnalata nel mese di luglio 2014 nel Parco del Ticino, in un'area ricadente tra le Regioni Lombardia e Piemonte. I competenti servizi fitosanitari regionali si sono prontamente attivati per condurre monitoraggi intensivi nelle aree colpite, sia sulle larve nel terreno che sugli adulti, al fine di definire l'estensione dell'infestazione e definire le misure fitosanitarie prioritarie da attuare. Sulla base dei dati di cattura delle trappole posizionate in tutta l'area, i predetti servizi hanno istituito ufficialmente una zona delimitata, costituita da una zona infestata e una zona cuscinetto circostante, ed avviata un'attività di divulgazione. Considerato l'elevato rischio fitosanitario, la problematica è stata più volte discussa anche nell'ambito del comitato fitosanitario nazionale, dove sono state identificate le misure fitosanitarie da adottare in via prioritaria per contrastare il diffondersi dell'insetto, e rappresentata in ambito europeo, in particolare al comitato fitosanitario permanente del 27 e 28 ottobre 2014. Pertanto, per rendere uniforme la disciplina su tutto il territorio nazionale e predisporre un monitoraggio molto capillare in tutte le Regioni, altresì predisposto uno specifico decreto ministeriale relativo alle misure fitosanitarie di emergenza, condiviso nel comitato fitosanitario nazionale che ha espresso il parere favorevole nella seduta del 24 febbraio 2016. Il decreto ministeriale è attualmente in corso di registrazione presso la Corte dei conti. Nello specifico, per le attività vivaistiche che ricadono nelle aree infestate, sono state previste disposizioni fitosanitarie per lo spostamento dei vegetali e dei tappeti erbosi, in modo da evitare il trasporto passivo di larve dell'insetto presenti nel terreno associato alle radici. Peraltro, per definire le modalità di intervento più idonee in relazione alle dimensioni delle popolazioni di insetto nelle varie aree, è stato concordato con le Regioni interessate l'istituzione di uno specifico gruppo di lavoro tecnico-scientifico a cui saranno presenti esperti, oltre che del Ministero delle politiche agricole, anche dei servizi fitosanitari regionali e del mondo accademico. Allo stato attuale, per le misure di supporto finanziario relative al contenimento dell'organismo nocivo, è possibile intervenire attraverso i piani di sviluppo rurale regionali, mediante interventi conformi all'articolo 18 del Regolamento UE n. 1305 del 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale In particolare, tra le tipologie di supporto che la misura può coprire, sono previsti, tra l'altro, gli investimenti per il ripristino del suolo agricolo e il potenziale produttivo di aree colpite da disastri naturali, condizioni climatiche avverse ed eventi catastrofici.

Pertanto, considerando che le aree colpite dal parassita rientrano nell'ambito delle aree naturali protette annoverate nella Rete Natura 2000, tali misure potrebbero essere applicate nel caso in esame.

polifago che si riproduce con una rapidità incredibile, come testimoniano i dati della Regione Piemonte, secondo cui sono si è passati da 26.000 esemplari adulti nel 2014 a ben 800 milioni nel 2015.

per quanto riguarda le politiche agricole, ad un assalto all'arma bianca di insetti che arrivano molto spesso da Paesi tropicali o che non sono autoctoni,

Nel condividere il sentimento di preoccupazione espresso dalla senatrice interrogante con l'atto in discussione, non può non manifestarsi in questa sede un sentito rincrescimento per gli episodi accaduti. accaduti. Per entrare nel merito delle questioni poste, si precisa che i due forti boati di cui è cenno nell'atto di sindacato ispettivo, avvertiti l'11 maggio 2015 in Valbelluna poco prima delle 10, possono essere ricondotti all'attività della missione con nominativo «Banshee», composta da due velivoli F16 statunitensi, appartenenti al 31° stormo Fighter Wing, di stanza ad Aviano. La missione, regolarmente programmata e autorizzata, prevedeva un volo di addestramento. La pianificazione della missione escludeva attività a velocità superiore a quella del suono e il suo profilo non prevedeva attività addestrativa a bassa quota. Durante tale volo, un velivolo statunitense ha involontariamente superato la soglia cosiddetta mach 1.0 in due occasioni. Il pilota all'atterraggio ha regolarmente segnalato l'avvenuto *bang* sonico alle autorità militari italiane e americane. In merito agli ulteriori aspetti evidenziati nell'atto, si rende noto che il traffico aereo operativo condotto a bassissima quota (BOAT) è specificamente regolato dalla direttiva «Regole del volo per il traffico aereo operativo» dello Stato maggiore dell'Aeronautica. Essa prevede, fra le altre prescrizioni, che i voli operativi devono evitare il sorvolo dei centri abitati tranne alcune eccezioni espressamente previste, quali, ad esempio, quelle per voli reali di difesa dello spazio aereo nazionale o esigenze di soccorso. Riguardo, invece, all'attività a velocità superiore a quella del suono, essa è disciplinata nell'annesso 6 della stessa direttiva, la quale chiarisce che deve essere effettuata sul territorio nazionale solo in specifiche aree e ad una quota non inferiore a circa 11.000 metri sul livello del mare e, comunque, non nell'area alpina. Inoltre, può essere effettuata solo di giorno (dalle 9 alle 20) e durante giorni feriali. I velivoli stranieri che operino all'interno dello spazio aereo italiano sono sottoposti alle stesse regole del volo dei velivoli nazionali ed è espressamente previsto che prima di condurre l'attività richiesta, debbano dimostrare di avere piena conoscenza delle procedure nazionali. In particolare, l'attività di velivoli degli Stati Uniti appartenenti a unità permanentemente stanziate in Italia - come nel caso di specie è regolata dal documento «Rapporti Italia-USA. Procedura operativa in materia di addestramento» del luglio 1997, emanato dallo Stato maggiore della Difesa, come perfezionato con protocollo successivo, in base al quale vennero individuate: nuove procedure per il volo a bassissima quota; a bassissima quota; la nomina della *US Authority* ad ogni base utilizzata dalle forze USA, responsabile dell'attività di volo e dell'adesione alle regolamentazioni italiane; venne creata la figura dei *liaison officer* nelle unità italiane e statunitensi per ottimizzare il flusso di informazioni; venne creata una *flight safety board* per incontri periodici sul tema della sicurezza volo (trattasi di periodici approfondimenti sul tema della sicurezza del volo organizzati dall'Aeronautica militare); vennero riviste le nuove procedure adottate al fine di assicurare che tutti i fattori pertinenti fossero considerati (rotte di addestramento, operazioni di volo degli elicotteri e dei velivoli ad ala fissa); vennero implementate nuove procedure all'interno dei vari accordi bilaterali e tecnici esistenti o da attuare in futuro. In ogni caso, con cadenza annuale, vengono sottoposte all'approvazione dei vertici militari nazionali le richieste addestrative dei reparti americani stanziati in Italia per l'anno successivo.

da parte del Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche, previsto dalla convenzione siglata nel febbraio 2010 tra il Dipartimento della pubblica sicurezza e l'Unicredit SpA. La convenzione con Unicredit è stata stipulata in attuazione del decreto legge n. 144 del 2005, che reca misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale e - in tale ambito - stabilisce che il Ministero dell'interno individui le infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale e provveda poi alla loro protezione. Alla convenzione con l'Unicredit ha fatto seguito nel marzo 2011 un analogo atto con il Gruppo bancario Intesa San Paolo. Entrambi gli accordi sono stati stipulati, oltre che su richiesta dei medesimi istituti di credito, anche sulla scorta delle indicazioni ricevute dalla Banca d'Italia, che le indicava quali "banche sistemiche", unitamente al gruppo Monte dei Paschi di Siena. I positivi risultati raggiunti in termini di sicurezza informatica hanno portato il Ministero dell'interno a proseguire la cooperazione con i due istituti bancari, tant'è che le convenzioni sono state rinnovate rispettivamente nei mesi di marzo e di aprile dello scorso anno. Va sottolineata l'importanza di tali tipi di protocolli, che agevolano sensibilmente il processo di allerta, la conseguente individuazione della minaccia terroristica o criminale e la successiva adozione delle contromisure, in quanto individuano a monte i soggetti idonei alla gestione di questo tipo di emergenze, fermo restando il monitoraggio ventiquattro ore su ventiquattro effettuato dal Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche. Con riferimento alla richiesta delle senatrici interroganti di stipulare le convenzioni in questione con la totalità degli istituti bancari italiani, faccio presente che, a legislazione vigente, la *ratio* di tali tipi di atti è quella di garantire la sicurezza di quei sistemi e servizi informatici che costituiscono infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale. Nell'atto di sindacato ispettivo sono richiamati due progetti che si pongono anch'essi l'obiettivo di una maggiore sicurezza delle transazioni e dei traffici informatici, ma da angoli visuali diversi da quello fin qui esaminato. Per quanto concerne il progetto di formazione "Occhio alla truff@: basta poco per navigare in sicurezza", faccio presente che l'iniziativa rientra in un più ampio contesto di campagne di prevenzione dei crimini informatici su Internet, promosse dalla polizia postale e delle comunicazioni a tutela degli utenti del *web*, in collaborazione con associazioni di consumatori, scuole, banche, università e altri enti. Invece, il progetto OF2CEN, citato dalle senatrici interroganti e nel cui ambito si collocano le convenzioni stipulate con Banca Sella e Carige, anch'esse menzionate nell'interrogazione, mira specificamente alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di criminalità informatica legati al furto d'identità digitale, in particolare nei servizi di *home banking* e monetica. Il progetto, finanziato dall'Unione europea e realizzato a livello nazionale grazie a un consorzio di organizzazioni del settore pubblico e privato, si è concretizzato nell'implementazione di una piattaforma informatica utilizzata per la condivisione di episodi criminali in danno dei clienti di servizi finanziari *on line*. Tra i *partner* dell'iniziativa figura l'Associazione bancaria italiana, che ha diffuso tra i suoi associati le modalità di partecipazione. Finora, le adesioni di istituti di credito e società emittenti carte di credito ammontano a una ventina circa e sono in continuo aumento. Il modello italiano di sinergia tra le istituzioni finanziarie e il Ministero dell'interno, realizzato con la piattaforma OF2CEN, ha trovato favorevole interesse anche in ambito europeo, tanto che sta per essere esportato nei Paesi dell'Unione europea; l'anno scorso il Dipartimento della pubblica sicurezza ha presentato un progetto per la sua estensione ai Paesi dell'Unione. Ritengo che le iniziative appena illustrate testimonino dell'elevato livello di attenzione che il Ministero dell'interno dedica al rafforzamento dei sistemi di controllo di quel "territorio virtuale" che è Internet; territorio dove un numero sempre maggiore di cittadini passa il proprio tempo - o meglio passa la propria vita - e dove quindi, al pari di quanto avviene nelle strade reali, si rende necessario garantire elevati *standard* di sicurezza che l'alta professionalità della polizia postale e delle comunicazioni riesce a garantire come testimoniato dagli apprezzamenti espressi in ogni sede da parte di operatori e di altre forze di polizia europee e occidentali. Signor Presidente, prendo atto della risposta ricevuta dal vice ministro Bubbico, per la quale mi ritengo soddisfatta per quanto riguarda l'impegno profuso al fine di garantire la sicurezza dei servizi e dei sistemi informatici delle banche

il più ampio possibile al fine di offrire alla maggioranza dei correntisti italiani la protezione e il monitoraggio del Centro nazionale anticrimine informatico, considerato che al momento - come da lei affermato - tali convenzioni sono state stipulate con due istituti di credito nazionale, quali Unicredit e gruppo Banca Intesa. Invito, ad ogni modo, il Governo e le istituzioni competenti a non sottovalutare l'importanza della prevenzione di ogni tipo di crimine, a maggior ragione di quelli informatici, al fine di garantire ai cittadini italiani degli *standard* di sicurezza

relativa all'efficienza delle misure di sicurezza all'interno degli aeroporti italiani e, in modo particolare, dell'aeroporto di Fiumicino, anche alla luce dei più elevati livelli di rischio a cui è esposta l'infrastruttura in relazione allo svolgimento del Giubileo della Misericordia. Va subito detto che, in base al Programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile, attuativo della normativa europea in materia, è il gestore di ciascuno scalo aeroportuale a dover redigere, attuare e mantenere aggiornato il programma per la sicurezza del singolo aeroporto. In tale ambito, il gestore è tenuto, tra l'altro, a garantire che il numero delle postazioni di controllo operative nell'arco della giornata sia costantemente proporzionato al numero dei passeggeri e che alla sala partenze accedano esclusivamente i passeggeri muniti di un idoneo e valido titolo di viaggio. D'altra parte, il vettore aereo ha la responsabilità di verificare al *gate*, all'atto dell'imbarco, la concordanza tra il nominativo del passeggero riportato nel titolo di viaggio e il documento d'identità dello stesso. Tanto detto e venendo all'episodio specificamente menzionato nell'interrogazione, informo che, effettivamente, il 6 settembre dello scorso anno un cittadino belga è salito a bordo di un volo Ryan Air con destinazione Bruxelles, in possesso di un idoneo documento d'identità e di una carta d'imbarco a lui intestata, ma avente una data diversa. Si trattava di un volo intra-Schengen, per il quale non sono previsti controlli documentali da parte della polizia di frontiera. Come da prassi, il personale del gestore aeroportuale ha sottoposto il passeggero ai controlli di sicurezza al varco Schengen T3. L'operazione è stata ripetuta al *gate* d'imbarco, ad opera del personale di terra del vettore. Sottolineo che, nella circostanza, entrambi i controlli sono stati effettuati manualmente, non essendo possibile in quel periodo effettuarli attraverso gli ordinari sistemi elettronici e di lettura ottica, danneggiati dall'incendio che aveva colpito lo scalo romano nel maggio 2015. Questi i fatti, dai quali si evince che alla base dell'episodio non vi è stato un errore di sistema, ma un errore umano, tra l'altro, non più ripetibile, atteso che nel frattempo i sistemi di controllo automatizzati sono stati ripristinati. In risposta ad altro quesito formulato dagli onorevoli interroganti, informo che, a partire dalla seconda metà dello scorso anno, il dispositivo di sicurezza aeroportuale relativo ai due aeroporti internazionali della Capitale è stato oggetto di un progressivo potenziamento, calibrato sui crescenti volumi del traffico passeggeri connessi allo svolgimento del Giubileo. Tale processo ha conosciuto un ulteriore impulso ed affinamento a seguito delle stragi di Parigi e di Bruxelles, del novembre 2015 e del marzo scorso e delle conseguenti analisi che sono state sviluppate in merito al *modus operandi* dei gruppi terroristici di matrice jihadista. In particolare, per quanto concerne l'aeroporto di Ciampino, è stata potenziata la sorveglianza delle biglietterie e della zona esterna, con l'impiego, lungo tutto l'arco delle ventiquattro ore, di personale del contingente militare dell'operazione Strade sicure, in aggiunta ai servizi espletati dalle forze di polizia dislocate nello scalo. Misure più articolate sono state adottate per l'aeroporto di Fiumicino, sul quale si concentra il maggior traffico nazionale ed internazionale di merci e di passeggeri. Anche in questo caso, si è puntato ad intensificare la vigilanza sulla zona biglietti e sull'area esterna, con l'impiego non soltanto del personale della polizia di frontiera e degli altri comandi delle forze di polizia operanti nell'aeroporto, ma anche di due ulteriori autopattuglie del reparto prevenzione crimine, nella fascia oraria diurna, e di una robusta aliquota del reparto mobile della Polizia di Stato durante la notte. Tali iniziative si aggiungono agli interventi che, grazie anche alle opere di ammodernamento dell'aerostazione avviate dopo l'incendio del 7 maggio 2015, mirano ad innalzare il livello complessivo di sicurezza, attraverso il miglioramento degli apparati tecnologici e l'adeguamento conseguente delle altre infrastrutture. In proposito, rappresento che il dispositivo dispiegato dalle forze di polizia può oggi giovarsi di un sistema di videosorveglianza con 2.000 telecamere, numero peraltro destinato a crescere ulteriormente entro la fine di quest'anno. Un altro settore su cui si è concentrata l'attenzione è la recinzione esterna dell'aerostazione, che, pur essendo già rispondente agli standard fissati dalle regolamentazioni comunitarie e dal programma nazionale di sicurezza, è stata irrobustita con opere di rafforzamento dei punti più esposti, compresi i cancelli di ingresso. Sono inoltre in corso gli interventi per migliorare l'individuazione rapida. In particolare, in aggiunta alle quarantacinque videocamere a circuito chiuso distribuite lungo il perimetro, capaci di coprire la fascia oraria diurna, è stata avviata la sperimentazione di un sistema antintrusione avanzato, con l'impiego di sette telecamere "ogni tempo", lungo un tratto di un chilometro particolarmente esposto. Nel contempo, è stato innalzato il livello della vigilanza del perimetro, che viene assicurata oggi non sono da due pattuglie itineranti di guardie giurate, incaricate dal gestore aeroportuale della protezione del patrimonio aziendale, ma anche da un servizio svolto lungo l'intero arco delle ventiquattro ore dal personale degli uffici e comandi delle forze di polizia operanti nell'aerostazione. A tali servizi, opportunamente integrati da aliquote della polizia di frontiera, si aggiungono le attività di vigilanza sulla fascia esterna dell'aeroporto, assicurate dal commissariato di pubblica sicurezza di Fiumicino. Questo assetto di sicurezza viene inoltre rafforzato dagli organi di polizia dislocati nell'aeroporto, anche con l'impiego di unità specializzate in occasione di voli sensibili e in tutte le situazioni di sospetta intrusione nella cosiddetta area operativa oppure ancora nei casi di tentativi di ingresso illegale sul territorio nazionale. Al dispositivo di sicurezza concorre anche il personale giurato incaricato dal gestore aeroportuale di controllare il possesso delle prescritte autorizzazioni da parte degli operatori e dei mezzi che circolano all'interno dell'area di volo. Anche gli aeromobili in sosta vengono continuamente vigilati da guardie giurate, le quali provvedono ad allertare le forze di polizia in presenza di anomalie o di eventi sospetti. Le misure appena descritte sono destinate ad un ulteriore affinamento, atteso che la prefettura di Roma sta coordinando le attività avviate nel gennaio scorso per il mirato aggiornamento dei piani di sicurezza Leonardo Da Vinci relativi agli scali di Fiumicino e Ciampino, con l'effettuazione anche di sopralluoghi *in situ*, uno dei quali si è svolto proprio nella giornata di ieri. Passando ora all'organico delle forze di polizia in forza all'aeroporto di Fiumicino, sottolineo che esso si compone complessivamente di 1.551 operatori, di cui 802 appartenenti alla Polizia di Stato, 103 militari all'Arma dei carabinieri e 646 unità alla Guardia di finanza. Di questo contingente, 440 unità compongono il dispositivo di sicurezza aeroportuale, costituito da aliquote di forze di polizia specializzate, affiancate da unità operative di pronto intervento, che utilizzano equipaggiamenti specifici e tecniche operative mutuate direttamente dai reparti speciali delle forze di polizia, i NOCS. Tale dotazione complessiva è il frutto anche di alcune assegnazioni dì personale disposte in connessione con l'evento giubilare. Di recente, infatti, il contingente della Guardia di finanza è stato incrementato di 104 unità, di cui 35 specializzate nell'antiterrorismo, mentre all'Ufficio di polizia di frontiera sono state assegnate ulteriori 25 unità. Quanto al diverso dimensionamento - riscontrato dagli onorevoli interroganti - degli attuali organici di polizia rispetto a quelli degli anni si ritiene che il dato vada letto alla luce della progressiva esternalizzazione di alcuni servizi di sicurezza e anche alle diverse responsabilità attribuite dalla legge all'operatore gestore dell'aeroporto. Al riguardo, evidenzio che con un decreto interministeriale risalente al 1999 sono stati devoluti ai privati i controlli di sicurezza dei passeggeri in partenza e transito, nonché dei bagagli a mano e da stiva. Nel medesimo senso, il decreto-legge n. 101 del 2013 ha previsto che, sotto la supervisione di un operatore di polizia, possano essere dati in concessione anche i controlli ai varchi *staff* e ai varchi carrai. E ancora, il Programma nazionale di sicurezza dell'aviazione civile ha previsto che, ai sensi del regolamento comunitario n. 185 del 2010, la vigilanza del sedime aeroportuale possa essere effettuata da guardie particolari giurate, sempre con la supervisione delle forze di polizia. In conclusione, alla luce delle articolate misure che ho appena esposto, ritengo di poter affermare che il dispositivo di sicurezza approntato negli aeroporti internazionali della Capitale sia adeguato a fronteggiare i rischi

Signor Vice Ministro, sicuramente esaustiva la risposta, in virtù del fatto che l'interrogazione è stata presentata l'8 settembre 2015, quindi prima dei tragici fatti di Parigi nonché di Bruxelles. un senso avvisare il Ministero dell'interno della situazione che si andava profilando e che purtroppo si è verificata, fortunatamente non in questa città (ma questo nulla toglie alla gravità dei fatti che si sono verificati nelle città europee). Quella situazione evidenziava aspetti che richiedevano un'attenzione maggiore da parte del Ministero, specialmente per quelli che erano i siti più sensibili, in questo caso l'aeroporto di Fiumicino.

non solo dei turisti, non solo di coloro che sono in transito, ma anche e doverosamente dei romani, soprattutto dei romani che vivono nelle periferie. Quindi, piuttosto che farle un'interrogazione, rubo questo minuto all'Assemblea per farle presente che nel frattempo a Roma stati, dal 2016: circa trenta denunce per aggressioni a danno del personale ATAC, un pestaggio su un autobus a Prati, un anziano scippato al Collatino, due turiste spagnole aggredite con un collo di bottiglie ad Ostiense, sala scommesse svaligiata a Pietralata, un cittadino albanese catturato a San Giovanni dopo un tentato furto e un altro al Casilino che ha tentato di violentare una prostituta. Poi, tanto per rimanere in tema, questa notte per non dover aspettare un altro anno, senza fare un'interrogazione - a La Rustica due persone sono riuscite a scassinare un bancomat con un carro attrezzi e a fuggire via con il bottino. allora, per avere messo in sicurezza l'aeroporto di Fiumicino, anche se un cittadino belga (oltretutto, visto quello che è accaduto, rendiamoci conto che cosa vive Roma ogni giorno),

Non vorrei che qualcuno dovesse rivolgere a questo Ministero un'ulteriore interrogazione perché vi rendiate conto che Roma sta attraversando sicuramente uno dei periodi più grigi della sua storia. Anche se nel centro storico avete messo ragazzi, più o meno ventenni, con un mitra in mano a presidiare quelle che secondo voi sono le zone più sensibili, continua a esserci una città che, nelle sue periferie, vive nell'insicurezza e nella paura.